Presidente, ieri il Centro della memoria di Cinisi, intitolato a Peppino Impastato e alla madre, ha subito un'ulteriore intimidazione mafiosa:

La memoria di Impastato è vivissima e nuoce ai criminali. I mafiosi devono avere la consapevolezza che non riusciranno a far tacere la memoria e già nei prossimi giorni la presenza del Presidente della Repubblica in Sicilia darà un chiaro segnale.

Grazie,

Come già previsto dall'ordine del giorno, oggi pomeriggio proseguiranno le votazioni sul disegno di legge relativo ai lavoratori stranieri clandestini e inizierà l'esame della delega sulla sicurezza sul lavoro. In relazione all'andamento dei lavori in Commissione, la discussione del decreto-legge sull'emergenza rifiuti in Campania potrà essere avviata nel corso della seduta antimeridiana di domani o, in ogni caso, a partire da domani pomeriggio. Pertanto, domani mattina potrebbe proseguire la trattazione della delega sulla sicurezza sul lavoro. Tenuto conto delle richieste avanzate da alcuni Gruppi, la ripartizione dei tempi per la discussione del decreto-legge è stata effettuata con opportuni aggiustamenti rispetto al criterio proporzionale. Restano poi confermati gli altri disegni di legge già previsti dal calendario corrente (delega liberalizzazione energia elettrica e gas; collegato servizi pubblici locali; legge comunitaria 2007), cui si aggiunge il disegno di legge recante norme fiscali per l'ammortamento di immobili e in materia di IVA sui veicoli. La ripartizione dei tempi, prevista dal Regolamento per il disegno di legge collegato e per la legge comunitaria, sarà definita dalla prossima Conferenza dei Capigruppo, nel corso della quale saranno altresì prese in considerazione ulteriori richieste di integrazione delcalendario avanzate dai Gruppi.

la gravissima situazione che si è venuta a creare all'Ospedale Sant'Anna di Ronciglione, dove è stato chiuso il reparto di ematologia, a seguito di tre decessi per il batterio *pseudomonas*. È una situazione grave, che ha determinato, ovviamente, il trasferimento di altri malati; grave soprattutto perché questo batterio, quando colpisce, provoca numerose vittime:

l'Ospedale. Purtroppo, non abbiamo trovato interlocutori in quanto non erano presenti né il direttore sanitario, né il direttore del reparto. non sia stato neppure avvisato il sindaco. Vogliamo sapere se sono stati osservati i protocolli, senza mettere naturalmente in discussione la professionalità

vi è stato un comportamento intollerabile da parte delle forze di polizia. È comprensibile che esse siano uscite da una certa tensione per le giornate di visita di Bush, ma non è tollerabile che nei confronti di queste persone, tra l'altro in età avanzata, vi sia stato un comportamento stigmatizzato anche dal suo successore Bonanni. Le chiedo, quindi, un intervento deciso per protestare e perché vengano presi i provvedimenti necessari, comprese le scuse ai pensionati, che meriterebbero, per le loro condizioni, un diverso trattamento da questo Parlamento e da questo Governo. **Sul calendario dei lavori

abbiamo dovuto - giocoforza - diluirlo, perché, stante il numero, ma soprattutto l'importanza, dei provvedimenti al nostro esame,

Grazie,

caratterizzati centralmente dall'intervento del Ministro dell'economia, che ha lanciato delle contestazioni specifiche alquanto gravi nei confronti del Comandante generale della Guardia di finanza. Queste contestazioni, secondo molti di noi (e credo anche secondo la stragrande maggioranza del Paese), costituiscono ed individuano fattispecie delittuose, di reato, ed io mi sono permesso, signor Presidente, di trasmetterle una nota, in data 8 giugno, che mi permetterei di leggere all'Assemblea, data la delicatezza del tema trattato ed anche per offrire ai nostri resoconti parlamentari il senso della nostra iniziativa e del nostro appello rivolto alla sua persona. Condivido e mi associo, tra l'altro, a quanto detto dal collega Castelli su quello che è stato, è e continuerà certamente ad essere il suo sforzo per fare in modo che durante la Conferenza dei Capigruppo si pervenga sempre a soluzioni condivise. Di questo le rendiamo merito, così come le abbiamo reso sempre merito del fatto di aver consentito a questa opposizione di godere di un diritto di parola ampio nei momenti in cui la politica del Paese postulava l'esigenza di confronti che si

Il Ministro dell'economia, nel rendere le comunicazioni del Governo sulla vicenda Speciale-Visco, non ha esitato a riversare specifiche accuse di rilievo penale nei confronti del generale Speciale e ciò senza fornire alcun concreto elemento di fatto che potesse in qualsivoglia modo sostenere la gravità del suo dire. In particolare, il Ministro dell'economia, dopo aver premesso di aver rilevato nell'agire del generale Speciale "gravi manchevolezze" sia sul piano dei "rapporti tra comandante della Guardia di finanza e potere politico" e sia su quello "dell'esercizio del comando all'interno del Corpo", ha accusato il generale Speciale:...»

dall'articolo 117 del Codice Militare di Pace II Ministro dell'Economia ha affermato: «... subito dopo che fra il comandante generale e il vice ministro Visco si erano definite le linee guida per gli avvicendamenti alla Guardia di finanza di Milano, il comandante generale interrompeva la procedura che lui stesso aveva iniziato comportandosi come se quella procedura non esistesse: di sua iniziativa e rompendo ogni comunicazione imboccava per proprio conto ed in segreto una strada del tutto imprevista». In altri termini, il Ministro In altri termini, il Ministro dell'Economia ha accusato specificatamente il generale Speciale di non avere portato a compimento l'incarico affidatogli dal vice ministro Visco, segnatamente quello di procedere agli avvicendamenti dei quattro alti ufficiali in servizio a Milano; e di aver disatteso l'incarico scientemente e senza ragione alcuna. Il che si inquadra nella richiamata fattispecie di cui all'articolo 117 del Codice militare di pace, secondo cui «il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione fino a tre anni». Evidentemente, stante la costante giurisprudenza della Suprema Corte e per il rispetto che si deve all'autonomia ed indipendenza della magistratura, tanto basta per investire della questione la competente autorità giudiziaria. Non è evidentemente questa la sede per specifiche elaborazioni giuridiche. Toccherà al generale Speciale, se lo vorrà, specificare che gli assetti normativi regolatori dei rapporti tra autorità politica e comandante generale della Guardia di Finanza non consentono incarichi del genere di quelli segnalati dal Ministro dell'Economia e che le procedure di trasferimento non sono proseguite in ragione dell'allarme lanciato ufficialmente dalla Procura di Milano con riguardo al grave danno che dai trasferimenti sarebbero derivati a delicatissime indagini in corso. Toccherà al Ministro dell'Economia, sempre se lo vorrà, specificare di essere incorso in un grave errore interpretativo della normativa esistente. 2) del reato p. e p. dagli articoli 110-656 C.p. Il Il Ministro dell'Economia ha affermato: «... Il 14 luglio veniva avviata in apparente consenso la procedura di trasferimento degli ufficiali di Milano; due giorni dopo, il 16, l'agenzia Ansa dava testualmente la seguente notizia: «UNIPOL, azzerati i vertici della Guardia di finanza in Lombardia partire da questo momento la stampa diventa il canale attraverso il quale filtrano tutte le vicende che riguardano il comandante generale mediante la pubblicazione di lettere e note ricevute o indirizzate alle autorità, compreso il Vice ministro ...Va detta qui una parola chiara sul preteso nesso tra il caso UNIPOL e questa vicenda. Contrariamente a quanto cerca di far credere una campagna di stampa in corso da circa un anno, il nesso manca di ogni riscontro ... La giusta autonomia del Comandante generale è degenerata in separatezza. Magistratura e stampa sono state, di volta in volta, usate per alterare il rapporto corretto con il Governo, per screditare l'Esecutivo, comunque per intralciarne il normale operato Mentre sulla scena ci si comporta in un modo, dietro le quinte si annodano rapporti con la magistratura e con la stampa». In altri termini, il Ministro dell'Economia, proprio nel riferire sulle presunte manchevolezze del generale Speciale, ha tracciato un quadro ricostruttivo in base ai quale è inevitabile addebitare all'alto ufficiale, in ragione degli asseriti anomali rapporti con la stampa, la responsabilità di aver veicolato all'Ansa la notizia di cui alla riportata nota di agenzia; quella secondo cui si stavano azzerando i vertici della Guardia di Finanza impegnati nel caso Unipol. Una notizia falsa, secondo l'opinione del Ministro. E, di certo, atta a turbare l'ordine pubblico in quanto tesa a sostenere l'ipotesi secondo la quale le autorità politica e militare avevano provveduto a trasferire taluni ufficiali della Guardia di Finanza solo perché impegnati in quelle indagini Unipol in cui apparivano esponenti di vertice dell'area politica di maggioranza. Anche in tal caso, stante la costante giurisprudenza della Suprema Corte e per il rispetto che si deve all'autonomia ed indipendenza della magistratura, tanto basta per investire della questione la competente autorità giudiziaria. Non è evidentemente questa la sede per specifiche elaborazioni giuridiche. Toccherà al generale Speciale, se lo vorrà, spiegare che non ha trasmesso alcuna notizia alla stampa in genere ed all'Ansa in particolare nonché che quegli ufficiali si erano interessati e/o si stavano interessando alla vicenda Unipol. Toccherà al Ministro dell'Economia, sempre se lo vorrà, addurre le prove in base alle quali ha affermato che il generale Speciale intratteneva anomali rapporti con la stampa, indicandolo nei fatti come la "talpa" della citata notizia Ansa. Toccherà sempre al Ministro dell'Economia, anche in tal caso sempre se lo vorrà, spiegare le ragioni per le quali, a fronte delle risultanze documentali di cui alle indagini Unipol, ha ritenuto di dover comunicare al Senato della Repubblica che nessun elemento lega e legava quei quattro ufficiali alla vicenda Unipol.

espresso riferimento alla scalata BNL come oggetto delle intercettazioni, quelle famose intercettazioni realizzate da quei vertici della Guardia di finanza. E la scalata BNL era una scalata fatta della compagnia UNIPOL.

«... tutta la vicenda è stata caratterizzata dall'assenza di una comunicazione serena e cooperativa, da mancanza di trasparenza, di prudenza, di riservatezza, oltre che da quel venir meno alle regole etiche e deontologiche che si chiama omissione una continua distorsione di regole e procedure ha finito per deformare l'autonomia, che è indubbia prerogativa del Corpo, in qualcosa di diverso che chiamerei separatezza, quasi che fosse venuto meno l'essenziale legame tra autorità di Governo e vertice del Corpo al servizio dello Stato II che equivale a dire che il Ministro dell'Economia ha accusato il generale Speciale di aver scientemente e reiteratamente violato la legge non consultando il Consiglio Superiore della Guardia di Finanza e ciò al chiaro scopo di avere completamente «le mani libere» nel portare avanti la sua gestione «personalistica» del Corpo, Non solo. Il che equivale a dire anche che il Ministro dell'Economia ha accusato il generale Speciale di aver conferito encomi ad ufficiali a lui «vicini» senza che ve ne fosse ragione alcuna, quindi con motivazione falsa, e ciò al chiaro scopo di favorirne la futura carriera per il peso che nella progressione hanno

un numero enorme di encomi solenni all'aiutante di campo, il quale, secondo l'opinione del Ministro scarsamente rispettosa dell'articolo 27 della Costituzione, Ometto alcuni passaggi, pregandola di poter allegare questa lettera alla copia del resoconto, perché possa essere trascritta nelle parti che ho omesso per rispetto nei confronti della Presidenza che mi invita a concludere. parte della lettera. «Per le argomentazioni sopra esposte ed in ragione del fatto che il pesantissimo atto di accusa da parte del Ministro dell'economia, contenente espressa denunzia di condotte configuranti ipotesi di reato, si è consumato nell'Aula del Senato della Repubblica, le chiedo formalmente, nella sua qualità di Presidente del Senato e per la sua conseguente responsabilità, di voler trasmettere copia del resoconto stenografico della seduta pomeridiana del 6 giugno alla procura della Repubblica di Roma, affinché, esperite la opportune indagini, voglia assumere le determinazioni di competenza nei confronti del generale Speciale, nonché, nel caso in cui dovesse procedere all'archiviazione delle accuse rivolte nei di lui confronti, per il più a praticarsi nei confronti di chi tali accuse non ha esitato a formulare. Alla procura della Repubblica di Roma ogni valutazione sulle affermazioni del Ministro dell'economia in merito all'asserita separatezza del Corpo della Guardia di finanza dallo Stato, della quale si sarebbe reso autore e protagonista il suo Comandante Generale con relativa catena di comando». Signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito questa lettura, chiedo che copia integrale della mia missiva possa essere allegata a questo resoconto, comprensiva delle parti che ho omesso di leggere e mi permetto di insistere in questa richiesta, data la delicatezza e la gravità dell'accaduto. Risponderò prestissimo alla sua lettera che mi era pervenuta, senatore Schifani.

ho una proposta sul calendario dei lavori sempre riferita a quanto è accaduto stamattina a Roma alla manifestazione dei pensionati. è stata, finita la manifestazione, un'azione di polizia assolutamente inaccettabile e sproporzionata rispetto al fatto che alcuni pensionati intendevano avvicinarsi a Palazzo Chigi per manifestare - giustamente è loro diritto - per un aumento dignitoso delle pensioni e per l'istituzione del fondo di assistenza.

pertanto che il ministro Amato venga a riferire in quest'Aula sul perché, il per come, la polizia ha assunto questo atteggiamento che giudico irresponsabile, inaccettabile e sproporzionato. *(Applausi

per segnalare che avevo chiesto a lei, come Presidente del Senato, e direttamente al Ministro dell'economia, di rendere noto all'Aula sulla base di quale atto formale l'attuale Ministro dell'economia esercita la delega sulla Guardia di finanza. Infatti, come risulta dagli atti, a tutt'oggi non esiste alcun provvedimento del Consiglio dei ministri e del Presidente del Consiglio dei ministri che deleghi sulla Guardia di finanza il Ministro dell'economia. Come ho detto non è un riassorbimento automatico perché il vice ministro Visco ha rimesso temporaneamente... PRESIDENTE. Questo con il calendario non ha nulla a che fare, senatore Baldassarri! A fine seduta le do la parola. Non possiamo andare avanti così! BALDASSARRI *(AN)*. Presidente Marini, il Ministro dell'economia non ha risposto in sede di replica. La prego di chiedere, come presidente del Senato, in base a quale atto il Ministro dell'economia ha svolto in quest'Aula

Il Ministro dell'economia, nella trasmissione «Speciale TG1» di domenica, ha riferito testualmente ciò che non ha riferito qui in Senato relativamente alla decisione del Consiglio dei ministri

e scopriamo che il Consiglio dei ministri partorisce idee senza che una testa le proponga - e non per mia proposta e capisco che possa essere criticata. Ora, questo rilievo era stato formulato da tutti i Presidenti dei Gruppi dell'opposizione durante le dichiarazioni di voto e il Ministro non lo ha detto. Capisco che il ministro Padova Schioppa, da grande tecnico, ha poca dimestichezza con la democrazia parlamentare, ma siccome è venuto a darci una lezioncina di chi comanda e di chi non comanda in democrazia, di chi decide e chi non decide, le chiedo formalmente, signor Presidente, che convochi al più presto il Ministro perché integri le mancate comunicazioni su cui abbiamo ahimè votato. *(Applausi

di legge Amato-Ferrero per il riordino generale delle norme sull'immigrazione, che verte sugli stessi argomenti (certo, anche su molti altri, ma pure su quello che stiamo trattando adesso). In Commissione - e poi anche in Aula - abbiamo assistito generico e non molto ben individuabile impegno del Governo a non esercitare la delega, una volta conferitagli dalla - io spero impossibile - approvazione del disegno di legge Amato‑Ferrero su questa disciplina che adesso stiamo trattando. Anche sulla base di ciò, in Commissione abbiamo avuto un atteggiamento collaborativo; poi, in Aula,

di varare, entro l'estate, un urgente decreto-legge estivo (così viene definito dall'agenzia di stampa) che estenda gli effetti dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione

come sia concepibile che il Governo, mentre il Parlamento sta esaminando - anche con una certa celerità - questo provvedimento, parli di varare un decreto-legge sull'identico argomento: è una cosa assolutamente inaccettabile

purtroppo - probabilmente verranno risolti sempre nel senso di allargare le maglie e cancellare i controlli. In questo modo, nel nostro Paese potranno venire - in primo luogo e, forse, anche esclusivamente - coloro che non vogliono rispettare le regole e poi,

Signor Presidente, anch'io, sulla scia di quello che diceva il senatore Malan, invito il Governo a chiarire, una volta per tutte, qual è il suo approccio al tema dell'immigrazione, perché fino a questo momento non vi è stato un disegno chiaro e coerente. Il primo atto di natura amministrativa e non legislativa è stato, poco dopo l'insediamento del Governo, il decreto flussi integrativo, che ha ampliato enormemente le possibilità di ingresso che erano state previste dal decreto flussi 2006, introducendo un principio che fa saltare in aria l'intero impianto del testo unico sull'immigrazione nella sua struttura originaria (quella cosiddetta Turco-Napolitano, risalente al che prevede una verifica attenta delle esigenze del mondo del lavoro, ma anche della capacità di assorbimento da parte degli enti territoriali rispetto ai nuovi ingressi regolari. Il principio introdotto con il decreto flussi integrativo è quello in base al quale ogni domanda presentata, al di là di come e da chi sia stata avanzata, deve trovare accoglimento, tant'è che lo scorso anno si fece un'operazione aritmetica: si calcolarono 520.000 domande presentate, si detrassero da questo numero complessivo le 170.000 che erano state previste con l'*iter* del decreto flussi originario e si consentì una riapertura dei termini, ma anche di possibilità di accoglimento di domande, di ulteriori 350.000 unità. Questo non è stato però l'unico provvedimento in materia. Recependo in termini di attuazione la direttiva europea 2003/86/CE, che non ha ricevuto un vaglio approfondito da parte delle Camere dal momento

inoltre, una proposta - l'Atto Camera n. 528, in questo momento in discussione nell'altro ramo del Parlamento - che introduce per lo straniero detenuto la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno o addirittura la carta di soggiorno in costanza di detenzione. All'interno di questo quadro (che è di natura amministrativa per i provvedimenti già adottati e di natura legislativa per quelli di cui si propone l'adozione) si inserisce un'enorme confusione, in termini di iniziativa del Governo, tra il disegno di legge legge in questo momento in discussione, quello che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile scorso e ciò che viene annunciato - lo ricordava prima il collega Malan - dal ministro Ferrero: un decreto‑legge che addirittura, azzerando il lavoro che il Senato, soprattutto in Commissione, ha svolto sul disegno di legge del quale ci stiamo occupando, immagina di tornare ad una dilatazione dell'articolo 18 dell'originaria versione del testo unico sull'immigrazione. In presenza di questa estrema confusione, credo che il Senato, che in questo momento esamina il disegno di legge sullo sfruttamento del lavoro degli extracomunitari, abbia necessità di comprendere in modo chiaro e coerente le intenzioni del Governo, di capire quali norme il Governo intende come prioritarie (e quindi da varare prima di ogni altra) e di comprendere se

Non abbiamo chiarezza su tutto questo e la attendiamo dal Governo anche per capire come orientare il nostro voto definitivo, oltre che sull'articolo 3 (sul quale sarà contrario, visto che c'è necessità di

spiegato in quale contesto normativo più generale queste norme si intendevano essere collocate. Nel corso della discussione, ho atteso più volte da parte del relatore, della maggioranza e del Governo

dal preannuncio - che sia il collega Malan, sia il collega Mantovano hanno ricordato - dell'intenzione, anzi ormai della decisione, del ministro Ferrero di presentare comunque un decreto-legge che ottenga risultati pressoché simili a quelli che si volevano ottenere, in un primo tempo, con la prima stesura del provvedimento Ora, se il nostro parziale favore a una discussione, a un dialogo e al tentativo di raggiungere un'intesa tra maggioranza e opposizione su questo disegno di legge nasceva dal fatto che la Commissione aveva messo riparo a molti dei palesi e gravi errori che il disegno di legge aveva nella sua formulazione originaria (proveniente dal Governo), è chiaro che l'annuncio del ministro Ferrero chiude la porta a qualunque dialogo e a qualunque interlocuzione. Ma c'è di più, signor Presidente. Oltre a lamentare il caos legislativo che il Governo sta introducendo, immettendo nel sistema delle imprese italiane un ulteriore livello di incertezza legislativa, che rende assolutamente problematico, a chi produce e a chi crea ricchezza in questo Paese, il farlo (e poi ci si stupisce che l'economia non procede), si aggiunge a questo un caos sul piano amministrativo, per quanto riguarda ciò che sta avvenendo nell'attuazione delle leggi oggi vigenti. vigenti. Non dimentichiamo che il disegno di legge del Governo di riforma dell'immigrazione tale è e resta e non può essere anticipato nella sua applicazione, visto che non ha passato il vaglio delle Camere. Ci si attenderebbe dal Governo, attraverso l'amministrazione, l'attuazione della legge vigente, che - ricordo ancora a tutti colleghi della maggioranza - continua ad essere la legge Bossi-Fini. Eppure, chiunque guardi nelle nostre città lo stato di applicazione della legge attualmente in vigore sull'immigrazione trova un allentamento che supera di gran lunga qualunque capacità interpretativa e spesso vìola palesemente la legge.

dall'attività delle forze dell'ordine, le quali ricevono direttive informali di agire come se la legge vigente non fosse tale. Su questo punto mi riservo di presentare interrogazioni con altri colleghi.

un quadro di caos legislativo e di legislazione a macchia di leopardo, occasione per occasione, di mancata risposta alle proposte che dall'opposizione, da parte di essa, da me e dal mio Gruppo erano venute

Personalmente ritengo che, per una maggioranza che ha fatto un *totem* del parlamentarismo, ciò sia veramente grottesco e in qualche modo ridicolo: più si è parlamentaristi a parole, più ci si

Allora, Presidente, siamo di fronte ancora una volta ad una iattanza, supponenza ed arroganza di un Esecutivo che, invece di confrontarsi di confrontarsi con una opposizione che ha aperto i lavori su questo disegno di legge con il massimo della disponibilità e della sensibilità - perchè noi siamo contro lo sfruttamento del lavoro

Vediamo, invece, che da altra parte si amano fare grida manzoniane, ma ci si disinteressa del tutto dell'attività legislativa ed il ministro Ferrero, invece di fare annunci in o di frequentare piazze deserte contro i nostri alleati, potrebbe più utilmente frequentare le Aule parlamentari, specie quelle dove forse è più difficile il cammino di certi provvedimenti per renderlo più agevoli, laddove l'opposizione tende la mano al Governo ed alla maggioranza ed invece si vede per tutta risposta quella mano morsa dalla iattanza del Governo. Dunque, rispetto a quanto avevo espresso in sede di discussione generale, è evidente che il nostro atteggiamento non può essere che di dura ed intransigente opposizione al provvedimento e questa è la prima occasione che abbiamo per dirlo con chiarezza. *(**Applausi del

Presidente, l'articolo 3 apparentemente tocca un aspetto di assoluta irrilevanza.

quella piccola legge che quel poco di buono aveva introdotto, cioè, di entrare almeno con un contratto di lavoro, cosìda «sfangare» lagiornata, da combinare pranzo, colazione e cena, senza dover pensare ad altro. Bene, arrivando tutte queste persone senza necessità di avere un lavoro, anzi, non potendo lavorare, perché qui si introducono norme severissime sul lavoro irregolare, ahimè saranno costrette a sbarcare il lunario in altra maniera.

Facendola breve, il grande ricco, dopo dieci giorni che si trovava in disgrazia, non sapendo e non essendo nemmeno abituato a vivere in mancanza dei minimi agi cui era abituato, si era ridotto non solo sulla strada, non solo

legge obbligheremo tutti gli immigrati che si trovano nel nostro territorio e che non sono regolari o a chiedere assistenza allo Stato o a mettersi nelle mani della criminalità, perché non troveranno più nessuno che neanche *pro* *bono* *pacis* gli potrà offrire una benché minima attività

le persone sulla strada della criminalità, perché la pancia bisogna riempirla, questo è un dato oggettivo, anzi è un dato fisiologico.

chi, una volta entrato sul territorio in modo irregolare, si metterà in mano alla criminalità organizzata, ma criminalizza coloro che, evitando di mettere in mano queste persone alla criminalità, danno loro un lavoro più o meno irregolare. Dal momento che qualcuno avrà anche consolidato questa posizione di irregolarità, si troverà nell'impossibilità di rispettare la legge,

di questo, non chiamiamolo datore di lavoro, ma offerente di merce di scambio. Bene, dal momento che il minimo preavviso è di otto giorni non si capisce perché una legge che va a criminalizzare colui che si trova in posizione critica deve prevedere un termine inferiore a otto giorni, al punto da fargli commettere un primo reato, perché mantiene un lavoratore in condizione non regolare, o un secondo reato, perché non gli consente neanche di dargli il preavviso minimo che sì dà a tutte le persone con le quali si interrompe un contratto contratto di lavoro. Per queste ragioni e per il fatto che non c'è veramente alcuna necessità di correre con questo provvedimento, crediamo sia giusto non approvare la formula, così come prevista nell'articolato, dell'immediata entrata in vigore della legge.

perché oggettivamente trovo questa disposizione assolutamente irragionevole, ma principalmente lesiva delle garanzie dei cittadini nel corretto rapporto che deve esservi

ma ha il senso di una «riconvenzione» delle disposizioni. Pertanto, interverrò, insieme ad altri colleghi, per dichiarare la mia posizione Senatore Ferrara, il riferimento è proprio ad emendamenti che presuppongono la presenza di un articolo. Quello in esame è un emendamento che non fa riferimento a nessun articolo, di una situazione assolutamente diversa e anche i precedenti che abbiamo vanno in questa direzione, del resto non capita spesso una simile situazione. Le do quindi la parola per dichiarazione di voto.

per motivi di urgenza - come detto dal relatore, dal Governo e dai senatori della maggioranza - una modifica al codice penale? Come si fa a spiegare un'urgenza con 22 parole di titolo? Ho l'impressione che il titolo sia, mi permettano i colleghi, leggermente

e poi, ancora, «lo sfruttamento dei lavoratori irregolarmente presenti». Vorrei capire perché è «grave» lo sfruttamento dell'attività lavorativa e non è invece «grave» lo sfruttamento dei lavoratori irregolarmente presenti:

in diversi aspetti e che comunque, proprio per l'utilizzazione di parole che non hanno più un significato, viene contraddetto nella sua efficacia dall'altro provvedimento che è al secondo punto dell'ordine del giorno. Signor Presidente, nel

Quale prova più evidente vi è del fatto che non soltanto il titolo, ma anche le disposizioni sono contraddittorie? Il titolo nella sua dizione è l'esemplificazione della contraddittorietà, della farraginosità e del pressappochismo

titolata della disparità e, quindi, dell'incostituzionalità del provvedimento. È il motivo per cui noi, oltre che essere contrari - come abbiamo dichiarato nelle ultime tre settimane - al provvedimento e favorevoli agli emendamenti che cercavano di correggerne gli errori, siamo anche contrari agli emendamenti che ne hanno appesantito le disposizioni e contrari non soltanto alle modifiche del testo, ma anche a tutto il titolo, così come è stato predisposto.

a riconsiderare il senso di questo intervento innovativo: disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa. Sono le stesse identiche parole che si trovano alla lettera Q del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge cosiddetto Ferrero-Amato: «favorire un'adeguata tutela delle vittime di riduzione in schiavitù», «delle vittime di violenza» o di «grave sfruttamento». Stiamo discutendo di una legge rispetto alla quale lo stesso Governo proponente ha adottato un'iniziativa più ampia che tra poco sarà portata all'esame del Parlamento. Non si riesce ancora a capire quale delle due iniziative sia preferita dal Governo. Nel frattempo un Parlamento, che certamente in questa legislatura non ha brillato per numeri di attività lavorativa e di produzione legislativa, rischia concretamente di realizzare un doppione. Coerente con questo titolo e egualmente non condivisibile è la parte conclusiva della relazione che accompagna il disegno di legge a firma dei due relatori Bianco e Livi Bacci. Scrivono nella relazione che si tratta di una proposta intesa a porre un argine a un fenomeno di grave degrado sociale, quale lo sfruttamento del lavoro irregolare associato all'intermediazione illecita di manodopera. Ma che cosa facilita questo sfruttamento, se non una presenza ancora più massiccia di stranieri che si trovano in posizione irregolare?

capire per quale motivo c'è un sfruttamento così diffuso e varrebbe la pena di chiedersi se ciò non dipenda anche da una presenza oltre ogni limite di irregolari, di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, presenza che è cresciuta negli ultimi 12 mesi e che si presume possa ulteriormente crescere a seguito di provvedimenti che si stanno varando o che sono stati appena varati. Vorrei ricordare, tra questi, una legge (approvata in via definitiva il 16 maggio dalla Camera con i voti contrari del centro-destra) che elimina la necessità del permesso di soggiorno per gli extracomunitari che intendono accedere in Italia per affari, turismo o studio per un periodo non superiore a tre mesi. mesi. La precedente normativa consentiva questo ingresso per un periodo massimo di tre mesi con un permesso di soggiorno che normalmente veniva definito turistico; le nuove norme, invece, permettono allo straniero, in questi casi, di limitarsi a dichiarare la propria presenza all'atto dell'ingresso al questore della Provincia nel cui territorio si troverà, per questo periodo limitato, l'extracomunitario. Tutti noi sappiamo che la gran parte degli stranieri irregolarmente presenti oggi in Italia sono tali non in quanto sbarcati clandestinamente sulle coste italiane, in modo particolare su quelle della Sicilia meridionale e di Lampedusa, ma perché sono entrati in modo regolare col permesso di soggiorno turistico e poi si sono trattenuti illegalmente oltre il novantesimo giorno. Se questo già è avvenuto in proporzioni consistenti (circa i tre quarti degli irregolari presenti in Italia sono tali perché hanno superato il termine dei 90 giorni dopo essere entrati con un permesso di soggiorno turistico), credo sia legittimo chiedersi quanti in più saranno presenti irregolarmente, avendo sostituito il Parlamento, su impulso o comunque con il consenso del Governo, il permesso di soggiorno turistico con una sorta di autocertificazione. È chiaro che, dilatandosi l'area della clandestinità, si dilati parallelamente l'area dello sfruttamento, perché il clandestino presente in Italia ha di fronte a sé la strada di cedere alla tentazione criminale o quella di lavorare, ma può farlo solo in nero perché regolarmente non può essere assunto con un contratto di lavoro. Sarebbe interessante anche capire se si intenda realmente dare un provvedimento di espulsione a quegli stranieri che sono stati liberati in virtù dell'indulto varato alla fine di luglio dello scorso anno

dicevo, oltre 10.000 extracomunitari clandestini sono stati liberati in virtù dell'ultimo provvedimento di indulto e non sono stati espulsi perché a loro è stato consegnato un foglietto con una semplice intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale.

di una norma penale, peraltro confusa - ci torneremo in sede di dichiarazione di voto conclusiva - e insufficiente a limitare e circoscrivere l'area del grave sfruttamento, quando quest'area è stata notevolmente dilatata da tutto ciò che è stato introdotto per via amministrativa o per via legislativa da questo Governo e da questa maggioranza negli ultimi dodici mesi.

si tradurrà, in virtù dell'articolo 6, in un incremento notevole degli stranieri presenti in Italia senza lavoro e quindi in una ulteriore facilitazione dello sfruttamento. L'articolo 6 del citato disegno di legge,

che in base al testo unico sull'immigrazione consentono il ricongiungimento familiare e quindi l'arrivo in Italia del coniuge o degli stretti familiari, a cominciare dai figli. Ciò significa che, in assenza di queste condizioni condizioni e di qualsiasi previsione temporale minima per realizzare il ricongiungimento, sarà possibile entrare in Italia sulla base della mera dichiarazione del convivente, che chiede di essere ricongiunto al proprio*partner* - con il quale non c'è neanche una convivenza di fatto perché si trova al di fuori dei confini nazionali - e ci si chiede poi questo *partner* come lavorerà. Quindi, si aumenterà la quantità di persone extracomunitarie che hanno necessità di lavorare e che, non trovandola, accederanno al lavoro in nero e quindi rientreranno nelle file dello sfruttamento. Allora, signor Presidente, non solo il titolo, ma l'intero provvedimento merita una sonora bocciatura.

provvedimento punitivo nei confronti di una certa parte della società italiana, quella che, per intenderci, voi non riconoscete dalla vostra parte e che in qualche modo condivide le vostre idee. In effetti, il discorso immigrazione andrebbe affrontato in maniera omogenea e complessiva e non con provvedimenti raffazzonati che vanno ognuno a interessarsi di un aspetto diverso senza mai avere in mente

rischiare di avere una somma di provvedimenti parziali che rendono ancor più confusa la situazione, di per sé, da un punto di vista ideologico, assolutamente non chiara. La Casa delle Libertà, invece, con il proprio provvedimento in tema di immigrazione, la cosiddetta che riprendeva le fila di un ragionamento portato avanti in malo modo dalla cosiddetta legge Turco-Napolitano, faceva rientrare il fenomeno migratorio in un fenomeno accettabile e gestibile, basato su princìpi condivisibili, oltre che presenti in tutti gli ordinamenti degli altri Paesi simili al nostro;

e, soprattutto, come possibilità di offrire adeguata assistenza, nel senso complessivo del termine, alle persone che arrivano, né di poter raccogliere, senza distruggerlo, il sistema socio-economico tradizionale

e, soprattutto, il rispetto delle quote; si partiva dal presupposto, ovvio e condivisibile, che nessun Paese può accogliere un numero illimitato di persone proveniente da altri Paesi. A maggior ragione, un Paese come il nostro che - per le osservazioni che ho appena evidenziato - ha una quantità enorme di limitazioni sia dimensionali che di capacità di ricchezza da distribuire.

proteggere le persone deboli che potrebbero cadere in una situazione di sfruttamento, ma finalizzata esclusivamente a punire i cittadini italiani che non sono dalla vostra parte. Peggio ancora se sono imprenditori o persone che magari fanno economia, fosse anche quella domestica della nonna del collega Divina, che comunque, avendo la possibilità di assumere una collaboratrice familiare, contribuisce in qualche modo al movimento economico del Paese. A voi non interessa se poi questa vostra legislazione aumenta il numero dei disperati che possono trovarsi in questa situazione; vi interessa solo punire le persone che fanno alcune cose. cose. Allora, in questo senso, c'è un altro ragionamento che si deve introdurre necessariamente: in base a quale principio costituzionale esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B? serie B? Adesso voi introducete di fatto questa fattispecie di cittadino, per cui se io sfrutto un cittadino italiano a tutti gli effetti commetto un reato minore, se sfrutto un cittadino extracomunitario irregolare

In base a quale principio costituzionale succedono cose del genere? Sarebbe come dire che se io vado a rubare in una banca di destra commetto un reato, se vado a rubare

e per il rispetto dei diritti dei cittadini, dovreste esserlo per principio nei confronti di qualunque cittadino o di qualunque persona. Se vogliamo approvare una legge inutile - perché ce n'è già una quantità industriale nel nostro ordinamento contro lo sfruttamento del lavoro nero o di qualunque altro tipo, va bene, ma sarebbe assolutamente inutile perché - ripeto - ce n'è già una quantità industriale nelle oltre 300.000 leggi che esistono nel Paese. Il motivo però per cui si elabora una legge che va a punire in maniera maniera particolarmente grave e pesante chi sfrutta quella categoria di persone, che voi peraltro con altre leggi incentivate a diventare sempre più numerose nel nostro Paese, oggettivamente mi sfugge. L'ho chiesto anche la settimana scorsa. Qualche settimana fa, forse qualche mese fa, da un'indagine si evinceva che i collaboratori dei parlamentari, circa 800-900 persone, erano nella stragrande maggioranza impiegati con un contratto in nero a 800-900 euro al mese. Come abbiamo detto in precedenza, siccome in questa legislatura più di 600 parlamentari sono di centro-sinistra, vuol dire che la gran parte di queste persone è alle vostre dipendenze. Allora vi pongo una domanda: perché un parlamentare che assume un laureato italiano a 800 euro al mese in nero è una persona rispettabile, mentre una persona anziana che in buona fede assume una badante - e magari commette una irregolarità formale e si accorge che questa badante, con un documento falso, è in realtà una clandestina - commette una colpa gravissima per cui può essere addirittura messa in carcere? Se questo è il vostro modo di vedere le cose e di amministrare il Paese, noi non possiamo assolutamente essere d'accordo. Peraltro, come abbiamo constatato qualche giorno fa, ormai anche la stragrande maggioranza dei cittadini non è altrettanto d'accordo con voi.

è stato profondamente modificato anche con l'apporto positivo dell'opposizione, tant'è che all'interno del dibattito in Commissione non erano state evidenziate

Stante la discussione generale, tutti i membri dell'opposizione presenti sia nella Commissione affari costituzionali

in quella realtà ed in quel settore della nostra economia, nei fatti, non può che esistere un grave sfruttamento del lavoro. lavoro. Al di là dei trattamenti economici, infatti, non vengono rispettate le disposizioni di legge, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, gli orari, la sicurezza e quant'altro. Inoltre, si prevede l'aumento

sociale. Per queste motivazioni, credo che il provvedimento risponda e cerchi di risolvere il problema, che sta diventando amplissimo

di lavoro minorile. All'interno di questa condizione, si colloca la condizione del lavoratore immigrato, sia esso clandestino irregolare che regolare.

alla sopravvivenza di questo fenomeno illegittimo che tutti diciamo di voler condannare. Il provvedimento cerca di affrontare e di risolvere anche questa particolare condizione, riconducendola ad alcune normative precedenti

di centinaia di migliaia di nostri lavoratori i quali, nel caso in cui questo disegno di legge, dopo essere approvato in questo ramo del Parlamento, verrà approvato anche alla Camera, si troveranno in una condizione di maggiore tutela, di maggiore rispetto

colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame riguarda un aspetto importante della problematica più ampia relativa alla presenza di stranieri irregolarmente presenti sul nostro territorio nazionale; problematica trattata da ultimo nel cosiddetto disegno di legge Amato-Ferrero, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile scorso, che sarà oggetto di approfondita discussione nei prossimi lavori parlamentari. Il disegno di legge che ci accingiamo a votare oggi contiene misure importanti per contrastare il fenomeno gravissimo dello sfruttamento della manodopera clandestina, misure valevoli tanto a legislazione vigente quanto nell'ottica della riforma complessiva della legge sull'immigrazione. Si tratta di misure necessarie per elevare l'attuale livello di civiltà che si registra nel nostro Paese, essenziali per ostacolare la prassi barbara del trarre profitto dall'impiego di lavoratori privi del del riconoscimento di ogni diritto, sottoposti in molti casi al ricatto per la loro presenza irregolare che li costringe a rimanere nell'anonimato. Anzitutto voglio sottolineare che la necessità di delineare strumenti concreti ed efficaci per il perseguimento della giustizia e dell'equità nell'impiego dei lavoratori stranieri sia sentita in egual modo da tutti i Gruppi politici, tanto che in Commissione si è arrivati positivamente alla formulazione di un testo nuovo rispetto a quello presentato dal Governo, che accoglie rilievi mossi anche dall'opposizione: ad esempio, quello di non modificare l'attuale formulazione dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, secondo il quale chi subisce violenza o grave sfruttamento potrà ottenere il permesso di soggiorno, qualora corra seri pericoli per la propria incolumità nel tentativo di sottrarsi ad una organizzazione criminale. Tuttavia, durante l'esame in Assemblea la sostanziale e proficua convergenza sul provvedimento

Sarebbe auspicabile che i Gruppi di opposizione riflettessero ulteriormente, convergendo su una valutazione complessivamente non contraria ad un provvedimento che mira al perseguimento di obiettivi fondamentali, quali sancire la punibilità penale (nuovo articolo 603-*bis* del codice penale) di una forma particolarmente feroce ed inaccettabile dello sfruttamento del lavoro irregolare, il cosiddetto caporalato, definire sanzioni ad esso correlate, che consistono nella reclusione da 3 a 8 anni, nonché nella multa di 9.000 euro per ogni persona reclutata e occupata, pena che aumenta se i suddetti soggetti sono minori o stranieri irregolarmente soggiornanti. Contro lo sfruttamento, e nell'ottica di regolarizzare il mercato del lavoro attraverso il ricorso a manodopera extracomunitaria regolare, anche la Commissione europea ha adottato, il 16 maggio scorso, una proposta di direttiva. prevede sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare, allo scopo di garantire che tutti gli Stati membri indistintamente introducano - ed applichino effettivamente - sanzioni analoghe. Il nostro Paese calcherà oggi il primo passo nella giusta direzione per combattere un fenomeno che lede gravemente i più elementari diritti dei lavoratori e che, inoltre, distorce il mercato del lavoro ed altera la reale concorrenza tra imprese. Per queste ragioni, annuncio a nome dei Popolari-Udeur il voto favorevole al provvedimento in oggetto. *(Applausi dei

negli interventi precedenti - si sia contrari ai princìpi espressi nel provvedimento stesso. Ovviamente siamo contrari a qualunque tipo di sfruttamento, sia nel lavoro che in qualunque altra attività o relazione umana, di un individuo

il fenomeno migratorio, soprattutto quello irregolare e clandestino, in maniera diversa da quello che è: un fenomeno che ovviamente al mondo esiste, che non bisogna ignorare, rispetto al quale ci si deve confrontare, ma che deve essere affrontato in maniera positiva e propositiva, all'interno di quelle che sono le possibilità effettive di accoglienza, di disponibilità di lavoro, di abitazione e di servizi che il Paese può dare. In questo senso, invece, il tutto si sta riducendo ad una demonizzazione, con fortissime penalizzazioni, nei confronti di chi mette in opera questo tipo di relazioni con persone

Ma estrarre solo questo aspetto della legge, per irrigidirlo ulteriormente, non ha nessun significato, se non - come dicevo prima quello di voler portare avanti un'impostazione ideologica del problema, che ormai, come si è visto, è largamente minoritaria nel Paese ed anche largamente minoritaria nei Paesi occidentali simili al nostro. Basta vedere quello che è successo negli ultimi mesi in Francia dove, dopo anni di delirio globalizzatore, in cui ognuno diceva di tutto e di più, quando è arrivata una persona con le idee chiare,

che la legge in vigore sanziona, ma sono situazioni che diventeranno sempre più frequenti nei prossimi anni se seguiremo la vostra deriva ideologica sulla questione. È chiaro che se l'immigrazione è gestita da una legge ragionevole,

lavoro. In un Paese normale fatti come questi non sono accettabili. Se il problema dell'immigrazione esiste, come esiste, lo si deve affrontare in manieraponderata, ragionando sui numeri, sui princìpi, sulle possibilità di effettivo inserimento. Oltretutto, non possiamo assolutamente condividere

cittadini italiani che, alla fine, avrebbero lavorato in Italia a 200 euro al mese come in Romania. Questo non sarebbe stato sfruttamento perché lo avrebbe fatto, in quel caso, uno dei vostri rappresentanti? Su tutto questo non avete niente da dire. Come non avete niente da dire, per esempio, sulle liberalizzazioni, per cui è bene che uno statale lavori trentacinque ore alla settimana, magari un po' meno, e faccia quattro mesi l'anno a casa, tra ferie, malattie e assenze non giustificate, mentre i barbieri, per tenere il passo con la concorrenza, devono lavorare sette giorni su sette, altrimenti chiudono bottega in favore dei loro colleghi Questo per voi non è sfruttamento?

colleghi, rappresentanti del Governo, il Gruppo della Sinistra democratica per il Socialismo europeo voterà a favore di questa norma per un insieme di ragioni. La legge Bossi-Fini, la normativa introdotta nella passata legislatura in tema di immigrazione, pur dichiarando di voler contrastare e limitare la presenza dell'immigrazione irregolare e combattere il fenomeno della clandestinità, lo ha di fatto alimentato. E nella clandestinità è tornato ad emergere ed è cresciuto in maniera drammatica il fenomeno del caporalato, lo sfruttamento dell'immigrazione

Una vergogna quella del caporalato che avevamo debellato, che pensavamo non dovesse più ripresentarsi nel nostro Paese e che dopo tanti e tanti anni è tornata nuovamente agli onori delle cronache ed è diventata uno degli incubi di tante campagne, di tante realtà. Ciò che hanno subìto tanti e tanti anni fa i nostri braccianti adesso è diventato l'incubo quotidiano di tanti lavoratori immigrati. Vorrei ricordare a quest'Aula alcuni passaggi

la circostanza che gli immigrati sono sottoposti anche a sfruttamento sessuale da parte dei loro datori di lavoro,

ad un ragazzo raggomitolato come un *peluche* sul pianale posteriore. Solo per questo trasporto, di soli dieci minuti, il caporale ha incassato 40 euro. Questa è la condizione quotidiana in cui si vive nelle nostre campagne, nel

cento non dispone di bagni e servizi igienici. La maggior parte dei lavoratori immigrati riesce a mangiare solo una volta al giorno, per lo più la sera, anche nelle giornate in cui lavorano nei campi per oltre dieci ore. cento dei lavoratori intervistati ha dichiarato di percepire meno di 25 euro per ogni giornata di lavoro. Molti riescono a trovare lavoro solo tre giorni a settimana e le loro entrate sono quindi molto ridotte.

cento degli intervistati ha dichiarato di avere subito qualche forma di violenza, abuso o maltrattamento negli ultimi sei mesi in Italia e nell'82 per cento dei casi, purtroppo, l'aggressore era un italiano. cento delle malattie diagnosticate è di origine infettiva, soprattutto patologie dermatologiche, parassiti intestinali, malattie del cavo orale e respiratorie. Queste sono le condizioni nelle quali sono stati condannati migliaia e migliaia

specificare meglio il reato di grave sfruttamento dell'attività lavorativa e offrire una *chance* alle vittime. È impressionante, signor Presidente e cari colleghi, l'atteggiamento contraddittorio della Casa delle Libertà. Questo provvedimento è stato approvato pressoché all'unanimità in Commissione, dopo essere

che all'epoca era Ministro dell'interno, in una delle sedute in cui si affrontava il tema dell'immigrazione, ricordò come

100 i casi di reati compiuti da immigrati regolari. È interesse quindi dell'Italia, è interesse del nostro Paese sconfiggere la clandestinità, dando la possibilità di una regolarizzazione, rompendo quel circolo vizioso che è stato alimentato in questi anni e che ha sospinto migliaia di persone, per necessità, a rifugiarsi nell'ingresso irregolare e nella clandestinità. è la necessità e il bisogno, invece, di fornire loro un'opportunità e un'occasione perché - ed è questo l'obiettivo ed il senso di questa norma e del nostro voto favorevole - dobbiamo in questo caso aiutare le vittime, aiutarle a denunciare i loro sfruttatori e colpire le organizzazioni criminali che si sono arricchite e si stanno arricchendo, ancora oggi, attraverso lo sfruttamento del lavoro nero, attraverso vere e proprie nuove forme di schiavismo. Per questo noi voteremo a favore di questo Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge, il cui testo è stato discusso nelle ultime sedute, intende promuovere l'adozione di nuove e più efficaci misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Non può certo sfuggire l'importanza etica, prima ancora che economica e sociale, che un simile disegno di legge riveste: concedere un permesso di soggiorno allo straniero che, sebbene presente sul territorio in via irregolare, venga sfruttato in forme ascrivibili ad una vera e propria schiavitù rappresenta un segnale di grande civiltà. Per questa via, inoltre, si va a colpire una grave patologia del sistema produttivo lo sfruttamento della forza lavoro, appunto - che non solo pone in essere situazioni gravemente lesive dei diritti fondamentali della persona, nei quali si riconosce la nostra tradizione culturale, ma contribuisce, in modo rilevante, anche a sostenere economie illegali e di matrice mafiosa che, in alcune parti d'Italia, sembra capace di descrivere zone franche e di extraterritorialità.

La lotta al lavoro nero e alle nuove schiavitù rappresenta un passaggio non più eludibile per la realizzazione di una società più giusta, più solidale e più inclusiva. Introdurre quindi fattispecie di reato per grave sfruttamento di manodopera rappresenta un'iniziativa del tutto condivisibile, che avrebbe dovuto incontrare la sensibilità del nostro partito ed il pieno appoggio dei nostri colleghi senatori. Tuttavia, è con profondo rammarico che mi vedo costretto a dichiarare il voto contrario del Gruppo dell'UDC ed essenzialmente per due ordini di motivi. Il primo consiste nella deriva ideologica che in qualche modo pervade il testo, sminuendone le nobili intenzioni ed anche il clima di collaborazione che, a tratti, era emerso in Commissione: una deriva ideologica che è ben palese in alcuni commi, meno in altri, ma che mette comunque ancora in evidenza una rappresentazione conflittuale del mondo del lavoro che, se mai sia esistita in Italia, oggi comunque appare del tutto obsoleta e superata. Il secondo motivo, non meno importante, riguarda il difficile coordinamento di quanto previsto da questo disegno di legge con la normativa vigente in tema di immigrazione. Sembra evidente che le norme che verranno introdotte possano provocare una sorta di sanatoria delle posizioni di decine di migliaia di lavoratori irregolari. Giova ricordare che la cosiddetta legge Bossi-Fini vincola la possibilità di entrare e continuare a risiedere in Italia ad un effettivo rapporto di lavoro, proprio per un motivo ben preciso, ovvero evitare che in Italia vi sia un gran numero di persone che si trovino in situazioni di soggezione e potenziale sfruttamento. La nostra preoccupazione è che, grazie a questa norma ed al suo meccanismo premiante, ci possa poi essere una corsa ad una sorta di «autodenuncia», ovvero all'uso di un giro di prestanome per arrivare alla regolarizzazione dei lavoratori sì sfruttati, ma comunque pur sempre clandestini, ovvero regolarmente presenti sul nostro territorio. Ora, un lavoratore sfruttato dal «caporale» è una persona costretta a vivere e lavorare in condizioni drammatiche e del tutto degradanti. Su questo non possono esserci dubbi. Ma tale lavoratore, sebbene sfruttato, è pur sempre una persona che si è introdotta illegalmente nel nostro territorio. Colpire duramente un crimine odioso come quello in esame, infatti, non può tuttavia portare ad avallare un comportamento come quello dell'immigrazione clandestina, che pur con tutte le giustificazioni del caso rimane, e deve rimanere, un comportamento da regolamentare e reprimere. Questo per ragioni, che a noi sembrano evidenti, di equità e giustizia non solo nei loro confronti, ma anche di quelli dei nostri concittadini, verso i quali non credo che questa Assemblea abbia minori responsabilità. Del resto, uno straniero che si trovi clandestinamente in Italia una volta ricevuto un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, come potrà mantenersi senza un lavoro? Potrebbe ben ricadere nella possibilità di essere di nuovo sfruttato, ovvero andare ad infoltire le fila della criminalità. Per tutti questi motivi addotti, il Gruppo dell'UDC non può che votare contro l'adozione di un simile disegno di legge.

Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà contro il disegno di legge al nostro esame a seguito della discussione che si è svolta in quest'Aula, delle perplessità sollevate che non hanno trovato risposta né da parte dei relatori, né da parte del Governo, di alcuni emendamenti che hanno peggiorato un testo che già sollevava molti problemi. Vorremmo condividere con la maggioranza e con il Governo una linea di prevenzione e di contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri. Vorremmo condividerla avendo presentato alcune proposte, anche in questa legislatura, che puntano a far luce sul fenomeno perché sia meglio conosciuto e perché si individuino gli strumenti più adeguati per affrontarlo.

ad un disegno di legge che ho presentato assieme a molti altri colleghi, che punta all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla condizione della donna extracomunitaria in Italia, che segue un *iter* molto rallentato ancora in Commissione.

rifiutare affermazioni come quelle che si sono ascoltate anche pochi minuti fa in quest'Aula, secondo le quali con la legge Bossi-Fini sarebbero aumentati i clandestini, diminuiti gli immigrati regolari e sarebbe stato reso più problematico il contrasto dell'irregolarità. È vero esattamente il contrario se si vuole far riferimento a dati oggettivi: il 31 gennaio di quest'anno una Commissione istituita presso il Ministero dell'interno, composta da funzionari del Viminale e da rappresentanti di organizzazioni che non fanno riferimento certamente né

Mistura, ha approvato un rapporto sull'attuazione del testo unico in materia di immigrazione in Italia. Facendo riferimento ai dati contenuti in quel rapporto, emerge l'esatto contrario di ciò che si è sostenuto in alcuni interventi provenienti dalla parte sinistra (in tutti i sensi) di questo Senato. È venuto fuori, per esempio, che mentre nel 2001 la stima dei clandestini presenti in Italia, formulata dal Dipartimento di pubblica sicurezza, era pari a 800.000 persone, al gennaio 2007 era pari a 300.000 è più o meno di ottocentomila? Sono aumentati o sono diminuiti, i clandestini? E nello stesso rapporto Staffan de Mistura si fa stato che, mentre nel 2001 gli immigrati presenti regolarmente in Italia erano un milione e mezzo, oggi sono oltre tre milioni e la differenza di un milione e mezzo è ampliamente superiore rispetto ai 650.000 regolarizzati negli anni 2002‑2003. Potrei dar conto - ma sarebbe troppo lungo farlo - delle operazioni svolte dalle forze di polizia, nel quinquennio passato, di contrasto nei confronti dello sfruttamento criminale della clandestinità; vorrei però conoscere i dati attuali, che purtroppo continuano ad essere poco noti. Mi chiedo il motivo per cui viene introdotta una norma, l'articolo 603*‑bis*, nel codice penale attorno a cui ruota questo disegno di legge. Nel nostro ordinamento forse non esistono disposizioni che puniscono chi impiega lavoratori stranieri clandestini? Basta fare una ricognizione elementare - qualcosa è riportato anche nel disegno di legge per convincersi del contrario: basta leggere, fra gli altri, l'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione. Forse non esistono norme che puniscono il grave sfruttamento con modalità di violenza o di intimidazione? Basta sfogliare il codice penale e consultare alcune leggi penali speciali per constatare il contrario. Esistono certamente nel territorio italiano situazioni di sfruttamento dei lavoratori stranieri anche gravi, ma l'esistenza di questo fenomeno, la sua consistenza, dipendono da un vuoto normativo normativo o piuttosto da un numero insufficiente di controlli riguardanti fatti che in alcune parti del territorio nazionale sono sotto gli occhi di tutti, fuorché di chi dovrebbe accertarli? È un problema di direttive, di risorse? Parliamone. Qualche giorno fa, intervenendo nell'altro ramo del Parlamento, il Ministro dell'interno ha confessato - senza però trarne alcuna conseguenza - di aver esortato i vigili del fuoco a non pagare più i canoni di locazione degli immobili nei quali sono allocati, perché la legge finanziaria (varata su impulso e su proposta del Governo di cui egli fa parte) ha tagliato pesantemente i fondi per il Viminale, nel suo insieme e in particolare per le Forze di polizia, e ha fornito anche alcune cifre sui debiti già maturati su questi tagli e sulle risorse in meno di cui si può disporre in quest'anno finanziario. Questo sarebbe un terreno di approfondimento e di confronto. Così come sarebbe interessante svolgere un confronto, anche con le organizzazioni sindacali, sindacali, relativo al ruolo del sindacato nel far emergere questo fenomeno nelle sue effettive dimensioni e risvolti qualitativi, al fine di prevenirlo e di combatterlo. Credo che tutti ricordiamo che il *leader* di un'importante forza sindacale, recatosi in quel di Foggia all'indomani dell'indagine giornalistica cui prima si faceva riferimento, fu molto critico, impietoso nei confronti dei responsabili locali del suo stesso sindacato, che, a suo avviso (ma se lo asseriva lui, doveva avere qualche ragione per farlo), non erano stati sufficientemente vigili nel far emergere il fenomeno a cui vuole far fronte questo disegno di legge. Appare veramente inaccettabile che, invece di dotarsi di strumenti operativi adeguati per applicare le norme vigenti, si inventi una norma nuova, assolutamente confusa e contraddittoria, che si aggiungerà a quelle già esistenti, ma non risolverà i problemi concreti di prevenzione e di contrasto. Non si può accettare la rinuncia a potenziare gli interventi concreti, la rinuncia a investire risorse, uomini e strumenti. Ci si sarebbe aspettati, dopo il grido di dolore del Ministro dell'interno di una decina di giorni fa, qualche provvedimento suppletivo rispetto alla legge finanziaria, qualche nota di variazioni di bilancio per colmare i vuoti finanziari che esistono sul fronte della sicurezza e del contrasto allo sfruttamento dei lavoratori: non c'è stato nulla di tutto questo. Si tacita la coscienza provando a fare la faccia feroce con una nuova norma incriminatrice. Verrebbe da dire al Governo che, se e di governare quindi anche questi aspetti della nostra vita sociale, forse qualche Sottosegretario in meno potrebbe far reperire risorse per mandare qualche ispettore del lavoro e qualche carabiniere in più per stroncare questi fenomeni. Domani forse ci si lamenterà della chiusura di qualche azienda per un mese, così come previsto da una pena accessoria introdotta con questo disegno di legge, per il grave sfruttamento di un solo lavoratore, magari sulla base di circostanze molto discutibili apprezzate dal giudicante. Concludo dicendo che riteniamo offensivo che dai banchi dell'attuale maggioranza si sostenga che la nostra opposizione a questo confuso disegno di legge sia segno di scarsa volontà di contrastare lo sfruttamento dei lavoratori stranieri. Il Governo di centro‑destra ha fatto emergere dal nero 650.000 lavoratori stranieri, dando loro non un timbro su un permesso di soggiorno, ma un contratto di lavoro, assistenza sanitaria e contributiva. Nel simbolo

ha ragione il senatore Mantovano: i nostri simboli fanno riferimento a una condizione del lavoro fatta di sfruttamento, anche dei minori, dei carusi sfruttati nelle zolfatare siciliane o delle mondine che hanno lasciato il segno nelle canzoni popolari delle campagne del Nord. Quei simboli parlano, però,

stato curioso, nel senso che il Governo aveva proposto un provvedimento per contrastare il fenomeno che le organizzazioni ufficiali americane chiamano lavoro forzato - quindi non una mia invenzione

A quel disegno di legge, che a mio avviso rispondeva bene alla necessità, abbiamo preferito in Commissione un altro percorso: confrontarsi tra maggioranza e opposizione per addivenire ad un testo che consegnasse al Paese una possibilità

dove il mercato criminale dell'organizzazione della riduzione al lavoro forzato incontra il mercato legale che per ciò stesso si nutre di quel mercato criminale, e, sostenendo il lavoro, sosteniamo anche la qualità dell'impresa e la necessità di qualificazione del nostro sistema di imprese. È una legge che ha contenuti europei; in tutta Europa si ragiona del contrasto al lavoro forzato e delle modalità del contrasto a tale lavoro. E non c'è nessuna ideologia in questo, se come ideologia s'intende una falsa coscienza; c'è, invece, una concezione del mondo che appunto riparta dalla condizione della civiltà del lavoro e dalla qualità dell'impresa.

È stato ricordato che oggi sui giornali è riportata un'inchiesta e una ricerca del CENSIS sullo sfruttamento dei minori, che parla di 400.000 lavoratori in età compresa fra i 7 e i 14 anni. che tale fenomeno è dovuto soprattutto ad un ambito familiare degradato che li avvia ad un inserimento in un contesto lavorativo degradante e di sfruttamento;

Grazie come era stato confezionato il provvedimento prima dell'esame in Commissione. Era un testo di disegno di legge - ripeto, di fonte governativa, e ciò ne aggrava naturalmente la rilevanza dei difetti che cercava di introdurre il reato di grave sfruttamento del lavoro, ricollegandolo, però, in maniera piuttosto semplicistica, arbitraria e direi anche piuttosto demagogica ad una modifica della legge Bossi‑Fini, in particolare ad una modifica dell'articolo 18 che prevede una fattispecie assai grave di sfruttamento del lavoratore extracomunitario clandestino, prevedendo anche un intervento di recupero, di assistenza o quant'altro.

parificato a quello, ripeto, dei soggetti sfruttati invece in situazioni di assoluto degrado, che comportava appunto questa parificazione: «previsione di «previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria». Questa era la «musica» del provvedimento, che poi collegava a questa modifica, già per di per sé grave e direi squilibrata della legge Bossi-Fini, la fattispecie penale del grave sfruttamento dell'attività lavorativa con sanzioni penali di assoluta rilevanza. Credo che l'opposizione nelle Commissioni riunite abbia svolto un lavoro estremamente costruttivo, perché non solo è riuscita a mettere in evidenza questa profonda contraddizione del provvedimento, ma anche a manifestare un intervento collaborativo (non è stato assolutamente ostruzionistico), tant'è che il provvedimento, alla fine, è stato in qualche modo rovesciato: cioè, la parte corposa del provvedimento è divenuta è divenuta la previsione della fattispecie della nuova figura criminosa, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, il «grave sfruttamento dell'attività lavorativa» che riguarda tutti i lavoratori, non solo gli extracomunitari ma anche i cittadini italiani e i lavoratori comunitari, con una fattispecie criminale assolutamente rigorosa, con sanzioni di assoluto rilievo proprio perché giustificate dalla gravità dei fatti previsti da questa norma, invece passare in secondo piano la modifica alla legge Bossi-Fini. Quali sono le critiche ancora attuali

per ragioni forse più ideologiche che di sostanza. È stato detto in quest'Aula dai miei colleghi che la legge Bossi-Fini è diventata per la maggioranza una sorta di idolo da abbattere. Posso capire che ci siano critiche, non è una legge perfetta, che ci possa essere la volontà di modificarla, però credo che, proprio per la delicatezza delle questioni che la legge ha affrontato e che si è cercato di risolvere attraverso una normativa quantomeno di sistema, occorra che si faccia un ragionamento di carattere generale, coerente nel proprio interno e con le parti della legge che dovessero restare invariate. Quindi, c'è un'occasione che questa maggioranza vuole vuole portare qui in Aula, cioè quella della riforma organica: ben venga questa iniziativa parlamentare; noi la verificheremo, la approfondiremo e potremo anche trarre gli elementi che guidano questa ulteriore riforma della legge sull'immigrazione. Invece la maggioranza cosa fa? Interviene sulla legge Bossi-Fini, che poi è la legge Turco-Napolitano corretta, con situazioni del tutto casuali, con opportunità del tutto casuali, una volta approfittando del recepimento della direttiva europea,

tratta di un metodo di lavoro che non possiamo condividere e non possiamo condividerlo nemmeno per questo provvedimento. Quindi, la nostra opposizione è forte soprattutto sulla seconda parte del disegno di legge in questione, che interviene in maniera estemporanea e non in maniera organica sulla legge Bossi-Fini. Vi sono però obiezioni che riguardano anche l'articolo 1, dove si prevede la norma penale principale, perché nei lavori di Aula vi sono stati almeno due emendamenti, dei non molti presentati, che hanno in qualche modo aggravato la situazione prevista dall'articolo 603-*bis* e hanno fatto venir meno o quantomeno hanno incrinato questo elemento di assoluta gravità collegato alla fattispecie penale,

e questo, dal punto di vista dell'applicazione della norma, è un elemento che può ridurre il rilievo rilievo criminale della fattispecie e quindi portare ad allargare l'applicazione della norma penale. Poi, alla lettera *c)* dello stesso comma 1, si è prevista la sospensione dell'attività dell'impresa, come pena accessoria, laddove si accerti l'occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante, mentre la previsione era di almeno tre

a danneggiare i lavoratori invece regolarmente occupati, così come si desume dal contesto della norma. Per queste ragioni,

*(Ulivo)*. Signor Presidente, colleghi senatori, colleghi del Governo, il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore di questo provvedimento. Esprimiamo un forte plauso al Governo per aver assunto questa iniziativa di particolare rilevo umano e sociale, nonché il nostro apprezzamento all'onorevole sottosegretario Marcella Lucidi, per l'impegno con il quale ha seguito l'*iter* del provvedimento; consentitemi di esprimere, inoltre, un ringraziamento ai colleghi relatori, Enzo Bianco e Massimo Livi Bacci, per la perizia con la quale hanno curato il lavoro nelle Commissioni e nell'Assemblea. Le norme di tutela dei lavoratori immigrati contenute nel provvedimento segnano una risposta efficace contro lo sfruttamento dei lavoratori regolarmente presenti sul nostro territorio e pongono un argine al vergognoso fenomeno del caporalato. Molti colleghi, di tutte le parti, hanno citato in quest'Aula l'inchiesta de «L'espresso», che riguardava la mia terra prima volta, fece conoscere al mondo intero episodi di grave sfruttamento dei lavoratori clandestini, ingaggiati dal caporale di turno, in molti casi legato alla criminalità.

e che dobbiamo cercare di sconfiggere. Svolse un intervento simile, tantissimi anni fa, un mio conterraneo, Peppino Di Vittorio, che ci insegnò che il caporalato era un triste fenomeno che doveva essere debellato. In realtà, esso è ritornato sotto altre sembianze e sotto altre spoglie: ecco perché il Governo e il Parlamento tutto hanno inteso hanno inteso presentare un disegno di legge contro lo sfruttamento dei lavoratori clandestini e contro il caporalato. Questo, colleghi, colpisce varie aree del nostro territorio e del nostro Paese, nonché diversi comparti produttivi, arrecando un grave danno al sistema economico

votate all'unanimità nelle due Commissioni riunite, quindi anche da un'opposizione che in quest'Aula ha poi scelto la strada incomprensibile dell'ostruzionismo e della chiusura dopo aver collaborato ad una rielaborazione del testo in Commissione e in Aula; lo stesso testo che è approdato in quest'Aula, che noi ci accingiamo a votare questa sera e che rappresenta, colleghi senatori, un contributo di elevata civiltà del nostro Paese del quale siamo fieri.

che punta a punire soprattutto la microimpresa, la piccola impresa. Questo è un Paese nel quale dilaga il lavoro nero; si dice che un terzo dell'economia italiana si regga sul nero, sul nero, che non sia emersa e che non si sa quando emergerà. Ma dal momento in cui in questo Paese dilaga il lavoro nero, come si fa a sostenere

nella disciplina sanzionatoria il sequestro dei luoghi di lavoro, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un mese? Come si fa a prevedere queste misure draconiane quando ci si trova di fronte al lavoro nero

Presidente, volevo già intervenire prima, all'inizio della seduta, per sottoporle un caso di questi giorni, quello di un giovane che ha perso la vita nel cercare di salvare dei bagnanti in Sicilia: Ivan Rossi, di Civita Castellana, città industriale della provincia di Viterbo. Questo giovane, alcuni giorni or sono, a Noto marina, in Sicilia, è deceduto nel tentativo di salvare la vita ad alcuni bagnanti in difficoltà: un mare che d'improvviso ha cercato l'atto eroico del giovane. Per alcune persone l'atto di Ivan è stato provvidenziale; egli però, ridotto allo stremo delle forze, non ha resistito allo sforzo. Il vescovo di Civita Castellana, monsignor Zadi, dice: «Ivan è stato definito un eroe (...) debbono ricordarlo e onorarlo per sempre. Non ci sono altre parole da dire, per tutti parla lui, con il suo esempio e la sua totale abnegazione verso il prossimo. Grazie Ivan». Questo giovane, con il suo gesto, ci fa riflettere, ci dimostra quanti di questi giovani hanno ben alti valori e sentimenti di altruismo, di abnegazione, di rispetto della vita. Invece, in altri casi, vediamo immagini martellanti, sulle televisioni pubbliche o private, di giovani che non hanno rispetto della cosa pubblica e offendono il nostro Paese con atti di violenza. Per questo ho avviato, insieme ad altri senatori e agli enti locali, la procedura per il riconoscimento al giovane Ivan Rossi dell'alto valore della medaglia d'oro al valore civile. A questo scopo, vorrei che quest'Aula del Parlamento, con un gesto che lascio a lei, signor Presidente, desse testimonianza ai genitori, ai familiari, agli amici, alla cittadinanza, al nostro Paese, del grande senso di rispetto per chi sacrifica la propria vita con altruismo, abnegazione e valore.

del direttore che è stato addirittura comandato dall'autorità che controlla l'ente stesso, rispetto ad una vicenda riguardante un comportamento antisindacale nei confronti di un dirigente sindacale,

Signor Presidente, lei ha già pronunciato la sua adesione come Presidente dell'Assemblea, quindi, non aggiungo altro se non condividere le parole del collega Giulio Marini perché questo ragazzo di Civita Castellana, in effetti, ha compiuto un gesto di grande generosità, di quella generosità di cui i giovani sono capaci, contrariamente alla *vulgata* che spesso li definisce incapaci di relazioni sociali e di sentimenti. Quindi, la sua sensibilità davvero può essere importante per dare un segnale da parte dell'Assemblea alla famiglia, ma anche a quella generazione di giovani che si comportano in questo modo. Grazie! Grazie!